link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 24 novembre. A partire dalla seduta pomeridiana di oggi proseguirà la discussione del disegno di legge su parchi e aree protette. In relazione ai tempi di trasmissione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti al provvedimento, l'ordine del giorno potrà proseguire con l'esame delle relazioni della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Il calendario della settimana è inoltre integrato con l'esame di ratifiche di accordi internazionali, in particolare l'accordo Italia-Francia sull'alta velocità, ove concluso dalla Commissione. La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito delle ratifiche, saranno discussi i disegni di legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario e sulla produzione vitivinicola, ove concluso dalla Commissione. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 16 novembre, alle ore 9,30, il Ministro degli affari esteri renderà un'informativa sulla situazione politica in Turchia. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti dei Gruppi per cinque minuti ciascuno. Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 novembre avrà luogo il *question time* con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il calendario della settimana dal 22 al 24 novembre prevede l'esame del decreto-legge sul sisma dell'agosto 2016 nonché - ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - del decreto-legge in materia fiscale. Restano confermate le mozioni già in calendario per le sedute di martedì 15 e 22 novembre. Infine, l'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 28 novembre al 2 dicembre.

interventi delle associazioni e lei, Presidente, le ha ricevute. Riteniamo assolutamente incredibile che non ci si voglia assumere la responsabilità di

si è arrivati comunque in Aula, tranquillamente, senza relatore. Per noi è una questione assolutamente prioritaria quindi chiediamo, ancora una volta, che

voteremo contro questa proposta di calendario. Siamo esterrefatti e allibiti dal continuo rinvio

e, in realtà, alla faccia della povera gente italiana e dei truffati! Sono in gioco miliardi di euro e non si intende far chiarezza al riguardo. E chi, se non il Parlamento, deve fare chiarezza? Si continua a rinviare. È un fatto inaccettabile, che non può essere ammesso in una democrazia vera e civile.

Grazie.

sia bene che l'Assemblea ne abbia contezza, perché si tratta di un problema molto importante che colpisce un po' tutti i Paesi occidentali (in particolare, europei). Il Governo britannico ritiene che la ipersensibilità ai farmaci possa diventare un problema devastante nel giro di pochi decenni e l'Italia è uno dei Paesi, se non il principale, in cui si usano più antibiotici. È pertanto importante trattare questo tema.

Grazie.

contrarre così i tempi della discussione di tre approfondimenti territoriali così differenti, in tempi così brevi, con una discussione generale unica svolta in anticipo sul previsto,

che seguono i nostri lavori e cui va tutta la nostra solidarietà e tutto l'impegno per poter avere le risorse per ricostruire le loro città.

il senatore Arrigoni aveva chiesto il differimento alla giornata di domani.

Il senatore Arrigoni può dare lettura del testo della mozione che ha firmato e la può illustrare

una per ognuna delle tre relazioni licenziate dalla Commissione d'inchiesta sugli ecoreati.

Le ho chiesto se sia emersa anche la terza relazione, quella sul sito di interesse nazionale di Bussi. Se così fosse, io ne sarei relatore, così come sono stato relatore nella Commissione d'inchiesta quando, diversi mesi fa, è stata licenziata Ho chiesto e chiedo ancora, signor Presidente, di avere un minimo di tempo e penso di interpretare anche il pensiero degli altri colleghi. Mi pare che la collega Nugnes si sia

le fasi di discussione generale e di dichiarazione di voto non devono assolutamente essere compresse, così come sono stati compressi i tempi quando, qualche mese fa, sono state trattate altre tre relazioni licenziate

Pertanto, un certo tempo ci sarà. Se lei comunque insiste nel volerla trattare in maniera disgiunta, votiamo sulla sua richiesta.

di un provvedimento importante e innovativo, che, per certi versi, può essere anche ulteriormente discusso, ma spero che la Camera dei deputati lasci lasci invariato il testo dopo una discussione che è stata molto lunga e articolata. Mi preme però sottolineare che è stato presentato un emendamento del relatore per l'istituzione di tre nuovi parchi nazionali, tra cui il parco del Matese. Esiste già il Parco regionale del Matese sul versante campano, ma non esiste quello sul versante molisano;

o emendamenti, l'istituzione di un Parco nazionale del Matese con le due Regioni, Campania e Molise, che vedrebbero così riconosciuta la tutela di un paesaggio straordinario

questa ipotesi di sviluppo come necessaria non solo per la nostra Regione, ma per l'intera Italia, perché abbiamo un patrimonio ambientale che non va

il benessere che può offrire un ambiente come il nostro, ma soprattutto per esaltare le filiere agroalimentari che fanno della nostra Italia e del *made in Italy* il vero traino del futuro del nostro Paese, sia sotto il profilo agricolo che sotto il profilo della trasformazione dei prodotti.

per poi trasmettere il testo alla Camera, che, a sua volta, possa approvarlo e licenziarlo nel testo approvato in Senato, perché la discussione è stata ampia. Di ciò va dato atto e merito al relatore e a tutti i componenti della Commissione, che hanno lavorato per realizzare un testo

Questa è la sintesi del direttore del WWF, Gaetano Benedetto, contenuta nel documento firmato da 17 associazioni ambientaliste che lanciano un grido di allarme per il disegno di legge di riforma

134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali e oltre 171 aree protette regionali; complessivamente parliamo di 870 aree naturali protette, di oltre 3.163 3.163 milioni di ettari terrestri e di 2,3 milioni di ettari di mare; di un giro d'affari di 2 miliardi di euro all'anno e di un fatturato di 9 miliardi; di 85.000 posti di lavoro, tra diretti e indiretti (il turismo naturalistico ha continuato a crescere nonostante la crisi). Inoltre, qual è il valore ecologico di questo immenso patrimonio? I boschi tutelati nei parchi italiani valgono, solo per la riduzione dei gas serra, quasi 600 milioni di dollari; un metro quadro di prateria di posidonia oceanica vale 2.244 euro all'anno in base alla produzione di ossigeno, all'assorbimento di carbonio e per la protezione delle coste dall'erosione. Tutto ciò avviene in parte grazie agli oltre venti anni di attuazione della legge n. 394 del 1991. Sicuramente non è una legge perfetta, ma ha rappresentato una storica battaglia, frutto di un dibattito culturale decennale sorretto da una filosofia della conservazione e protezione dei valori ecologici. la legge ha venticinque anni e nel 1991 non c'erano la Convenzione internazionale sulla biodiversità, né la Strategia nazionale per la biodiversità, né Rete Natura 2000, né la Convenzione europea del paesaggio, quindi occorreva una revisione.

noi piuttosto sintetizziamo con semplificazione (che per voi significa mancanza dei dovuti controlli), valorizzazione (ossia mercificazione in evidente conflitto d'interessi), politicizzazione e territorializzazione a discapito della competenza e della specializzazione in tutela e conservazione della biodiversità. (ISPRA) assume un ruolo più rilevante, ma ancora una volta in assenza di nuovi oneri per lo Stato, ossia ancora una volta si attribuiscono nuove mansioni senza i dovuti sostegni finanziari.

Entra a gamba tesa Federparchi, che assume la titolarità di rappresentanza istituzionale degli enti gestori delle aree protette (un monopolio della rappresentanza degli enti gestori), sebbene Federparchi non sia un'associazione di categoria che riunisca tutti i soggetti che hanno oggi la responsabilità della gestione. Si tratta di un fatto né giustificato né corretto. In pratica, il consiglio direttivo si sbilancia tutto sulla rappresentanza politica, territoriale e imprenditoriale, a discapito della competenza scientifica e della salvaguardia della biodiversità. L'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 specificava in maniera inequivocabile che i componenti del consiglio direttivo sono individuati tutti tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette

Oggi, volontariamente, si cambia. Si specifica infatti che i componenti del consiglio sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura (in maniera generica), oppure nella gestione delle aree protette (che è un'altra cosa), oppure tra i rappresentanti della comunità del parco (ossia politici), secondo le seguenti modalità: il 50 per cento dei componenti su designazione della comunità del parco (sindaci e presidenti di Regione), specificando che almeno due dovranno

è un burocrate che, se pure esce dall'anacronistico albo dei direttori, non si delinea per competenze specifiche nel settore della salvaguardia, come dovrebbe. Si voleva addirittura, in una prima versione del testo, che questa figura perdesse la sua indipendenza e che fosse nominato direttamente dal presidente: questo ci dice molto sulla filosofia generale che ha dettato la riforma. Nel regolamento del parco interviene il silenzio-assenso del Ministero dell'ambiente e della Regione. Nel procedimento di approvazione del piano è acquisito il parere vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (una novità è vero), ma poi interviene l'atto unico autorizzativo che include anche la domanda di autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nel parco, che viene attribuita all'Ente parco, facendo fuori di fatto La fase di valutazione ambientale degli enti preposti la si inserisce nella definizione degli obiettivi, a monte, ma la si esclude dall'effettiva fase di controllo dei progetti, che si andranno a realizzare a valle. Il diniego del nulla osta dell'Ente parco è immediatamente impugnabile: è scritto nero su bianco. La filosofia della mercificazione parte dal finanziamento dei parchi attraverso le *royalty*. È assurdo il previsto meccanismo di pagamento agli enti di *royalty* da parte dei titolari di attività economica di elevato impatto ambientale, seppure già esistenti. In una prima fase del testo non era specificato o meglio non non era posto questo limite: è stata una modifica del relatore in Commissione. Chi ci dice che un emendamento in futuro non interverrà a modificare questo limite, visto che questa è la filosofia? Comunque, il rischio di gravi condizionamenti dell'operato dell'ente è senza dubbio già elevatissimo ora nella valutazione dei soli casi di rinnovi, estensioni o ampliamenti delle concessioni, seppure esistenti. All'ingresso i visitatori probabilmente dovranno pagare il biglietto. Sì prevedono anche proventi dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta, che, come per le *royalty* e per tutti quei sistemi di autofinanziamento che vanno in dirittura di collisione con gli interessi della salvaguardia, ci appare grave. Si tratta di un disincentivo persino al controllo che si dichiara di voler realizzare all'introduzione illegale di specie alloctone. Si potranno anche avere pericolosi effetti collaterali con la modifica proposta della normativa sulla caccia, che potrebbe portare anche ad un avvio di procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. [**Presidenza del vice Quindi, mentre da un lato si vieta esplicitamente la caccia in un articolo specifico, con artifici si apre alla caccia, con la giustificazione della necessità del controllo della fauna selvatica. È però già stato dimostrato, in altre parti, che queste non sono soluzioni valide e risolutive del problema e anzi alimentano il circolo il circolo vizioso del mercato illegale dell'inserimento di specie alloctone e distanziano dalla meta dell'eradicazione. Per sostenere economicamente i parchi abbiamo anche la concessione onerosa del marchio, che non ci appare certamente una maggiore garanzia di qualità, anch'esso in evidente conflitto di interesse con gli obiettivi. Viene introdotta, all'articolo 26, una delega al Governo per l'introduzione dei sistemi volontari di pagamento dei servizi ecosistemici.

delega al Governo non ci rasserena, nei termini dei possibili aumenti tariffari che ricadrebbero sull'utenza né nella valutazione disinteressata dell'opportunità di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune.

siamo arrivati, forse, alla conclusione della prima fase del lungo *iter* di approvazione del disegno di legge che propone interventi di modifica della disciplina sulle aree protette nazionali anche con riferimento alle aree marine. Il primo esame di uno dei disegni di legge in materia risale addirittura al 2013, ma oggi dovremmo essere giunti alla mediazione di un nuovo e più completo testo, tutto volto alla valorizzazione di queste aree, anche mediante una definizione e una distinzione tra parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali, cui si affiancano anche le aree marine protette. Le aree protette rappresentano, infatti, un patrimonio nazionale ambientale di notevole importanza: la moderna nozione di "bella Italia", che è di natura estetica e culturale, non può prescindere dalla consapevolezza di essere eredi e custodi di un ingente patrimonio naturalistico, che contribuisce alla formazione del concetto di "specifico italiano". quasi in ogni Regione troviamo zone di meravigliosa bellezza, che come tali devono essere valorizzate in ossequio al principio di compatibilità tra ecosistemi naturali e attività antropiche, sociali ed economiche. L'Italia - con con i suoi quasi 3 milioni di ettari di superficie a terra, e altrettanti a mare, tra aree naturali protette, parchi nazionali, riserve naturali statali, aree naturali marine protette, parchi sommersi il santuario dei cetacei, parchi naturali e riserve naturali regionali - è uno dei Paesi che negli ultimi dieci anni ha dato il maggior contributo in Europa allo sviluppo di un sistema di aree protette, passando dal 3 per cento ad oltre il 10 per cento di territorio tutelato. Tutti auspichiamo pertanto che questo patrimonio si possa convertire in un'opportunità di sviluppo sostenibile, date le enormi potenzialità di ricettività turistica di cui dispongono queste aree che - ricordiamolo - contengono ecosistemi prevalentemente o largamente intatti, ambienti e paesaggi di un rilievo tale da richiedere un intervento istituzionale per garantirne la conservazione alle future generazioni. Si è perciò reso necessario questo adeguamento della normativa, al fine di integrare e modificare la legge quadro del 6 dicembre 1991, n. 394, che in alcune sue parti appare oggi abbondantemente superata. Il compito del legislatore è stato, quindi, quello di bilanciare la protezione e la conservazione delle biodiversità, che trovano nelle aree protette un argine decisivo alla progressiva estinzione di un numero sempre maggiore di specie animali e vegetali, con la loro naturale vocazione allo sviluppo, comprensivo delle opportunità economiche che ne derivano, in un quadro di compatibilità e adattamento alle esigenze di tutela ambientale.

Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Putignano, in provincia di Bari, in cui è già operante l'oasi di protezione faunistica del Barsento istituita nel 1976 con atto della Regione Puglia. La perimetrazione del parco coincide con la detta oasi di protezione faunistica e ne amplia il territorio di competenza. La valenza naturalistica, paesaggistica, storico-archeologico-architettonica del territorio ricadente nella perimetrazione effettuata a suo tempo dalla Regione Puglia è nettamente testimoniata dall'unicità fisica e ambientale. Una parte dei Comuni ricadenti nell'area - come Noci e Alberobello - ha provveduto da tempo a sancire nei consigli comunali l'adesione al parco, approvandone i confini. Per questi motivi, sicuramente ricorrono le condizioni per adottare azioni di tutela, salvaguardia e difesa degli equilibri naturali del territorio individuato, nonché di valorizzazione intesa come fruizione ecosostenibile delle molteplici emergenze culturali rappresentate dalle doline, dal sistema di grotte e ipogei, dai sentieri, dal patrimonio boschivo a base di lecci e roverella, dalle storiche masserie, dalle diffuse architetture in pietra a secco caratterizzate soprattutto dalla presenza di trulli, dalle aziende agricole a vocazione di allevamento bovino ed equino. Pressoché al centro dell'area individuata insiste la basilica altomedievale di Barsento, con valenze storico-archeologiche che datano all'età del ferro. Ho cercato perciò di perorare questa causa attraverso un emendamento e un ordine del giorno, che garantiscano il riconoscimento di questa zona come Parco nazionale del Barsento, favorendo così la possibilità di incrementare le risorse finanziarie, umane e strumentali, utili a realizzare gli interventi

che ho presentato il primo giorno di apertura di questa legislatura, nello stesso testo approvato nella scorsa legislatura proprio qui al Senato, e che pertanto, anche su mia richiesta, nel settembre 2013,

Va bene, ci può anche stare; nell'utilizzo dilatato e sicuramente opzionale dei calendari del Parlamento italiano questo ci può anche stare, però adesso finalmente lo stiamo esaminando.

osservo con piacere è stata mantenuta - in ordine alla concezione delle aree protette, della loro funzione sul territorio nazionale e soprattutto sull'economia e sullo sviluppo socioeconomico del Paese. Questa legge era nata ventidue anni fa per

per la protezione di aree che non sono solamente ambientali. Vorrei infatti ricordare ad alcuni colleghi che mi hanno preceduto, e a chi segue questa vicenda, che il territorio italiano ha italiano ha pochissimi centimetri quadrati di natura vergine, ma ha migliaia di chilometri quadrati di aree che sono rilevanti dal punto di vista ambientale per effetto antropologico, cioè per l'intervento dell'uomo.

da parte dell'uomo in senso positivo, continuasse e che dopo un periodo di conflittualità, ripeto, tra estremisti della protezione ambientale ed estremisti della speculazione, ritornasse ad essere anch'essa una saggia e precisa

il senso dell'estetica e il senso dello sviluppo, come si è detto, sostenibile, o forse, come io ho sempre detto durante questi dibattiti, della sostenibilità dello sviluppo, più che dello sviluppo sostenibile. In quest'ottica si inquadra sicuramente questa riforma che tardava da anni e che salutiamo con piacere. Non sarà perfetta, ma vede un maggior coinvolgimento degli enti locali e quindi una maggiore integrazione tra enti locali

andando a pescare nelle speculazioni di loro convenienza. Infatti non sono speculatori solamente alcuni personaggi di cui naturalmente non condivido l'attività

con diffidenza la presenza degli Enti parco perché temevano non solo la conflittualità sull'attribuzione dei poteri ma anche, spesso, la conflittualità relativa alle soluzioni per il territorio. nella *governance* degli Enti parco di attività di categorie come gli agricoltori, che sono sempre state ritenute nemiche della conservazione dell'ambiente e che invece è dimostrato, soprattutto dai dissesti idrogeologici che colpiscono le zone più marginali del Paese, che sono essenziali

anche come secondo lavoro in un'ottica non di profitto ma di conservazione di un bene che magari hanno acquistato con fatica, impiegando le risorse provenienti dal loro lavoro. Se non inserissimo nell'ambito della *governance* dei territori i rappresentanti di queste categorie, continueremmo ad avere conflittualità che non giovano, abbandono di molte terre e conseguenti disastri idrogeologici dovuti anche a questo. Non solo, continueremmo ad avere anche l'invasione delle specie alloctone, con gravi danni non solo per l'agricoltura, ma anche per la biodiversità. I cosiddetti integralisti dell'ambientalismo, che ripopolarono indiscriminatamente boschi e foreste con razze alloctone, come il cinghiale carpatico, oggi piangono la scomparsa del cinghiale italiano e la devastazione della stessa biodiversità.

Una sfida che deve essere risolta anche dagli enti locali, mettendo al governo dei parchi gente che ne capisca (e mi si perdoni la semplicità dell'espressione), che non travalichi il proprio incarico per interessi particolari, ma che abbia riguardo ad un interesse specifico dell'ambiente. In questo bisogna anche considerare che lo sviluppo e il mantenimento di vastissime aree (sono state ricordate le cifre dell'enorme incidenza delle aree protette nel nostro Paese) dipende anche dagli uomini che le abitano, cioè dall'incentivazione del ripopolamento

e chi è demandato alla protezione dell'ambiente e, quindi, anche l'abbattimento delle barriere di diffidenza che finora sono esistite tra Comuni ed Enti parco. Un abbattimento anche di alcune prerogative riservate alla casta, quella sì, di associazioni che hanno ritenuto di poter fare il bello e il cattivo tempo, passando spesso sui piedi degli operatori economici, degli agricoltori, degli operatori turistici e anche, in alcuni casi,

a Carrara, al monte Amiata e a tutto ciò che il mondo ci invidia e che noi oggi, giustamente, vogliamo tutelare. Ma non possiamo tutelare stabilendo che una macchina per l'estrazione del marmo non entra più in quel territorio, perché rovineremmo completamente il significato di quell'ambiente, che evoca scenari danteschi, che evoca Michelangelo e tutto ciò che è connaturato alla nostra cultura e che può anche essere connaturato ad aspetti del nostro futuro.

fase dell'esame degli emendamenti potremo cercare di ottenere, non nel senso politico del termine, ma dal punto di vista della nostra prospettiva, il cambiamento di alcuni aspetti che, punto di vista, sono un po' aberranti, soprattutto in alcuni sistemi penalizzanti di piccoli operatori economici. Certamente, però, siamo soddisfatti

provvedimento introduce una meccanismo nuovo, perché non istituisce un vero e proprio parco nazionale, ma chiede al Governo di definire un'intesa fra due Regioni che ora gestiscono i due parchi regionali, la cui unione definirà la nuova area protetta unitaria.

testualmente, che «il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto». Quindi - ci tengo a precisarlo - l'atto legislativo in esame non lede in alcun modo l'autonomia del Veneto e dell'Emilia-Romagna, che peraltro hanno contribuito alla stesura di questo articolo. Ci sono pochi dubbi sull'opportunità di istituire un'area protetta unitaria del Delta del Po, con un'estensione maggiore del 50 per cento rispetto al celebre Parco della Camargue, paragonabile ai grandi parchi del delta del Danubio. un'area protetta con 400 specie animali autoctone fra uccelli, molluschi, pesci, anfibi, rettili e mammiferi, che nel 2015 è stata riconosciuta come unitaria riserva di biosfera Si tratta, quindi, di un delicato ecosistema sostanzialmente unitario, pur nelle ovvie differenze legate all'ampia estensione e alle complesse vicende storiche e amministrative. L'opportunità di istituire un ente unitario è legata anche alla convergenza di tutta l'area - realizzatasi nel corso degli ultimi anni - verso la vocazione turistica ecosostenibile e verso attività economiche ecocompatibili. L'unificazione di questa grande area protetta va nella giusta direzione amministrativa, ossia quella di far corrispondere la geografia di un ente gestore con l'effettiva unitarietà geografica e socioeconomica di un territorio. Ciò accade ogniqualvolta vi è coraggio di superare visioni localistiche, ad esempio quando i Comuni mettono insieme le loro funzioni o addirittura procedono a fusioni, con grandi benefici per i cittadini, di breve e anche lungo periodo. Del resto, già grandi aree protette italiane insistono sui territori di più Regioni, pur mantenendo una gestione unitaria. Nel caso del nuovo Parco del Delta del Po, l'unificazione della gestione eviterà contraddizioni e diseconomie di scala, mentre l'attività di programmazione potrà godere di maggior respiro. non va trascurato il grande vantaggio di *marketing* implicito nell'assumere un'immagine unitaria per tutta l'area protetta. Tutto ciò avverrà - lo ribadisco - senza mortificare in alcun modo l'autonomia delle Regioni interessate, né tantomeno gli interessi delle comunità locali.

ad esempio, ai ragionamenti che faceva prima il senatore D'Alì riguardo al coinvolgimento degli enti locali o dei soggetti che sono all'interno dei parchi. Ritengo che sia un passo in avanti

valutazione riguardo all'importanza e alla valenza dell'istituzione di un parco naturale, di un'area protetta o di un'area marina protetta e sostanza. Si è sempre di più consolidato il concetto che intorno a un parco e con l'istituzione di un parco innanzitutto si realizza un'importante opera di educazione nei confronti di chi vive in un certo territorio, soprattutto delle nuove generazioni; sia per quanto riguarda l'approccio e il rapporto con la natura, sia per quanto riguarda il rispetto di principi come quello di legalità e di tutela di certi territori, di certi

Oltre a questo, cioè all'ovvio concetto della prevenzione che consegue all'istituzione di un parco naturale,

che stava dietro all'istituzione di un parco, con il Ministero dell'ambiente che, con un suo decreto, congela, blocca, vincola e quindi affligge il il territorio oggetto di quell'intervento. Oggi invece dobbiamo passare più decisamente ad una logica premiale: il parco come vantaggio, come un'operazione che desta un interesse non solo economico, ma certamente un interesse importante per il territorio, che condivide e non subisce più quel parco. Questa secondo me è la chiave interpretativa più moderna, che

Ora, a me sta a cuore un altro problema all'interno di questa discussione, che poi consegue all'approvazione di questo provvedimento, rispetto alla quale - come ha già detto il collega Liuzzi - esprimiamo una valutazione favorevole.

la cosa più importante è quello che succede il giorno dopo l'approvazione, cioè come vogliamo istituire nuovi parchi e come vogliamo far funzionare i parchi che già esistono e con quali risorse. Abbiamo notato che uno dei problemi, soprattutto negli ultimi anni, è stata la mancanza di risorse, la mancanza di risorse, che ha portato il Ministero e gli enti locali, che credevano in queste operazioni, ad arrendersi spesso (direi quasi sempre) anche di fronte a territori che invece chiedevano a gran voce l'istituzione di

anni sono tantissimi, sono molti di più dei tre anni di cui parlava il senatore D'Alì per fare approdare la legge in quest'Aula, e sono trascorsi sostanzialmente inutilmente

per condurre e concludere gli studi necessari per la perimetrazione ed emanare il decreto di istituzione, ma soprattutto, poi, per far funzionare, dal giorno successivo, l'area marina protetta.

della Regione Puglia, che avevano emanato atti deliberativi e avevano impegnato somme, così come indicato e richiesto dal Ministero. Non possiamo più

alla Penisola italiana per le esigenze del territorio italiano, per essere stati un *hub* per gli immigrati fino a qualche anno fa, almeno fino agli inizi del 2000, in modo cospicuo (e ancora continua un servizio

infrastrutture importanti; penso a elettrodotti o a gasdotti che si ipotizzano, in alcuni casi, o addirittura si realizzano, in altri. Ebbene, una forma di risarcimento in questo senso dovrebbe essere riconosciuta; non si tratta di dare soldi, perché nessuno chiede soldi. Si chiede l'istituzione di un'area marina protetta. Devo ringraziare il relatore, che ha voluto ben delimitare, con un proprio emendamento, l'area, così come era stata, più o meno, richiesta dai territori interessati, che assumerà il nome di Capo d'Otranto, Grotte Zinzulusa e Romanelli. Chiedo al Governo e al Sottosegretario qui presente di fare uno sforzo ulteriore, il giorno dopo l'approvazione in Assemblea di questo provvedimento, con il prossimo treno della manovra di bilancio, per dare la giusta considerazione a quei territori che non chiedono infrastrutture inutili, ma che chiedono soprattutto di tutelare il proprio *habitat* naturale e di poterlo fare in una chiave moderna, intelligente e con grande sensibilità.

era necessario un intervento normativo che valutasse l'esperienza di questi anni e l'aggiornasse alla luce delle nuove emergenze ambientali e delle direttive comunitarie, che nel frattempo hanno dettato agli Stati membri sempre più puntuali incombenze in tema di siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale. Ricordiamo, infatti, come le principali criticità che sono state rilevate, a proposito di aree protette, riguardassero la mancanza di chiarezza normativa, la scarsa disponibilità di risorse finanziarie, il riconoscimento completo del ruolo di istituzione territoriale a ogni effetto, l'assenza di programmi nazionali di coordinamento e sostegno. Per le aree marine protette si eccepiva la mancanza di un organismo uniforme di gestione e di norme chiare, nonché la carenza di una relazione organica con le rispettive gestioni a terra e, inoltre, l'assenza di risorse predefinite. Allo stato attuale in Italia esistono più di mille aree protette che, in termini di estensione, rappresentano più dell'11 per cento del territorio italiano. Alla legge n. 394 del 1991 siamo certamente debitori per la costituzione di un sistema forte di conservazione di una biodiversità eccezionale e la potenzialità della valorizzazione della stessa a fini socioeconomici compatibili. Questi elementi, in molte aree protette - purtroppo non in tutte hanno inciso sullo sviluppo locale e favorito la partecipazione delle popolazioni e la democrazia, diventando fattore di crescita civile e culturale, oltre che di recupero di identità territoriali. la necessità di un'ulteriore crescita del modello di sistema, di un'ulteriore spinta e di un contagio delle gestioni virtuose con altre che lo sono state in misura minore in questi anni. Era, quindi, necessario un intervento del Parlamento per mettere mano

per estendere la gestione nello specchio d'acqua prospiciente dei parchi nazionali che si affacciano a mare, e della definizione «di valore naturalistico ed ambientale» ai parchi naturali naturali regionali. Inoltre, si disciplinano appositamente le aree marine protette, ponendo fine a quelle deleterie discrasie che molto spesso vedono due enti gestori differenti per le aree marine protette e per i parchi terrestri.

e non rendono un buon servizio nemmeno alle finalità istitutive dell'area da proteggere. In questo senso, quindi, ben vengano la razionalizzazione della gestione e il contenimento dei costi, ma anche l'appianamento dei potenziali conflitti tra enti gestori diversi e vicini. È altresì importante che la gestione dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) ricadenti in un parco naturale nazionale o regionale sia di competenza del corrispondente ente gestore. E ciò significherà che le valutazioni di impatto ambientale saranno rese dallo stesso ente gestore del parco naturale, che non potrà che giovare allo snellimento delle procedure burocratiche, eliminando duplicazioni di valutazione e contenendo i tempi per il rilascio dei necessari pareri. Ci preme sottolineare l'importanza che l'istituzione di un nuovo parco assorba tutte le aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso. A ISPRA sono attribuite le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientale e di ricerca, in materia di biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Per quanto riguarda gli organi di gestione dell'Ente parco, sparisce la «giunta esecutiva» del parco. Ciò gioverà certamente non solo ai costi, ma anche alla celerità delle decisioni. Vengono meglio definite e aggiornate le funzioni del presidente del parco, cui spetta la fissazione degli obiettivi e l'effettuazione della verifica in merito alla realizzazione degli stessi, esercitando anche le funzioni di indirizzo. Ancora, nel segno del contenimento dei costi e della celerità dei lavori, va la previsione del taglio del numero dei componenti del consiglio direttivo, che scende da 12 componenti, come previsto della legge del 1991, a 6 componenti, oppure a 8, a seconda della dimensione territoriale del parco. Un discorso un po' più puntuale merita il concetto di «aree esterne» o «aree contigue» ai parchi e alle riserve, richiamato in più punti dal testo, che non ha mancato di suscitare qualche perplessità e necessità di approfondimento, se non altro terminologico. Ricordiamo, infatti, come il concetto di aree contigue abbia rappresentato una novità introdotta proprio dalla legge quadro sulle aree protette. Infatti, attorno ad alcuni parchi nazionali e regionali preesistenti alla legge n. 394 del 1991, erano state istituite zone di pre-parco, viste come zone "cuscinetto" fra l'area protetta e il restante territorio, concepite come zone di naturale espansione della medesima area protetta, ma di aree contigue non vi era traccia. Probabilmente il concetto di aree contigue o aree esterne al territorio protetto è nato da un conflitto - potremmo dire - ideologico, dell'atavico contrasto tra mondo venatorio e mondo animalista. In realtà, si è visto che, dal punto di vista dell'esercizio della caccia, ha avuto scarsa rilevanza, mentre rischia di incidere in modo notevole su tutti gli altri aspetti di gestione del territorio. Per questa ragione l'aggettivo "contiguo", che significa situato nelle immediate vicinanze, adiacente, rischia di essere investito da un problema di insufficiente chiarezza, perché lasciato in balia di un'alea di interpretazione eccessivamente variabile e non fornisce sufficiente certezza, nemmeno quando è messo in relazione funzionale con la conservazione

non costituisce area protetta e, quindi, non è soggetta all'ingerenza gestionale dell'Ente parco, salvo alcuni poteri specifici, nel concreto non sono mancati casi di conflitto con gli enti territoriali, che si sono sentiti vulnerati nelle loro competenze ordinarie di pianificazione del territorio esterno al parco. Probabilmente si dovrebbe insistere di più nell'impegno di creare più sinergie tra enti gestori, Comuni e Regioni per creare più intese, al fine di avere ben presente che gli *habitat* naturali sono un valore fondamentale per la sopravvivenza della nostra stessa specie da governare con equilibrio e saggezza. testo in esame rappresenta certamente una riforma necessaria del sistema di tutela delle aree protette. La lunghezza dell'*iter* è giustificata dal gran tempo che è stato necessario per mettere in evidenza le luci e le ombre del sistema vigente, nonché le criticità e anche le nuove aspettative dei territori. Dobbiamo certamente proseguire nello sforzo di conservazione degli ambienti naturali, non tanto perché siamo obbligati a farlo dalle direttive europee più avanzate, ma come esigenza culturale e di stile di vita di tutti noi uomini. Nel far questo, comunque, non dobbiamo dimenticare che le aree protette devono superare il livello base del puro e semplice conservazionismo, per fare un vero salto nel terreno delle opportunità di sviluppo dei territori protetti, che hanno tutte le caratteristiche per essere accolte nella sensibilità di chi vi abita e opera come una risorsa in grado di apportare benessere, sviluppo, occupazione e ricchezza nel segno della sostenibilità e dell'equilibrio.

che individuava i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette. Oggi si sente l'esigenza di rivedere quel testo per andare incontro al mutato contesto e per garantire agli enti di gestione, in base all'esperienza acquisita, un coordinamento migliore e più efficiente. Il disegno di legge che esaminiamo oggi ha proprio questa ambizione. Al tempo stesso, però, è sempre più evidente come la difesa della biodiversità e della natura si debba accompagnare sempre più alla valorizzazione di un capitale naturale che assume diverse dimensioni. Ne sono esempi il turismo ambientale, le produzioni agroalimentari tipiche di qualità e la valorizzazione del territorio. Tuttavia, per comprendere a pieno la presente proposta, bisogna ricordare che già la legge n. 394 del 1991, nella sua originaria versione, è servita a costruire un sistema un sistema integrato di aree protette, nazionali e regionali, grazie alle quali nel nostro Paese si sono attuate politiche di conservazione della biodiversità fino ad allora impensabili. Tutto questo non va ridimensionato, ma va trasformato in un modello basato su buone pratiche da allargare a quelle zone di territorio italiano che sono uniche per il contesto paesaggistico e di biodiversità che rappresentano. Non mi soffermo certo a fare una analisi dell'articolato, già esaustivamente compiuta dal relatore, pur tuttavia non mi sottraggo dall'esporre alcune mie considerazioni sulla bontà del provvedimento. Innanzitutto, la sfida di oggi - e il presente disegno di legge, a mio giudizio, sembra averla compresa bene - non è solo la conservazione della natura, ma anche la sua valorizzazione.La rete dei parchi e delle aree protette del nostro Paese è un volano economico e occupazionale, soprattutto nell'agroalimentare e nel turismo sostenibile. Una natura tutelata e valorizzata, infatti, garantisce una qualità della vita sana: quello tra ambiente e agricoltura è dunque un binomio imprescindibile. Inoltre, i numerosi turisti *ecofriendly* che ogni anno frequentano i parchi e i territori vicini costituiscono un valore economico, come confermano diversi rapporti sull'attrattività e la qualità della vita di dette zone. Quindi, creare e supportare soluzioni innovative che collegano la conoscenza e la tutela della biodiversità alla promozione dei territori e delle eccellenze agroalimentari è non solo un dovere per noi in quanto legislatori, ma anche un'opportunità economica e sociale. Approfitto dell'occasione, poi, per rimarcare che bisogna puntare sul rinnovamento del sistema di *governance*: una gestione istituzionale condivisa e più vicina ai territori, più adeguata all'ottica della nuova visione di economia circolare

sia stato il frutto di una mediazione con tutti i soggetti interessati, dalle associazioni ambientaliste a quelle di categoria, agli enti e alle comunità locali. Nel testo che stiamo approvando, poi, sono confluite gran parte delle istanze proposte da tutti i Gruppi presenti in Commissione: una prassi positiva che vale la pena sottolineare. Gli aspetti maggiormente innovativi sono presenti in norme diverse, come la maggiore valorizzazione dei siti di Rete Natura 2000, l'attribuzione di una maggiore importanza al piano del parco (che assorbe principi e norme dei piani paesaggistici), ma anche in deleghe importanti come quella per la nascita del Parco del Delta del Po, Po, prima illustrato dal collega Dalla Zuanna. Infine, un'altra importante innovazione è rappresentata dalla norma secondo cui le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali. Per queste motivi, volendo fare un ragionamento d'insieme, penso che, unitamente alla legge sugli ecoreati, al collegato ambientale e al riordino dell'ISPRA e del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente, il presente provvedimento sia una delle riforme in campo ambientale che stanno caratterizzando positivamente questa legislatura. Non di meno, il disegno di legge contiene misure che, a completamento delle prescrizioni comunitarie, tengono assieme tutte quelle sensibilità che favoriscono la completa valorizzazione delle aree protette italiane. Infatti, a livello europeo la direttiva Habitat indica le finalità di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli *habitat* naturali. Concludendo, signora Presidente, l'occasione che ci viene data con l'approvazione di questo provvedimento non solo riguarda gli aspetti ambientali, ma significa anche affrontare con mezzi adeguati sfide nuove come il cambiamento climatico e la trasformazione degli *habitat*: solo così l'Italia potrà valorizzare al meglio valori storici, culturali e antropologici peculiari propri del suo territorio.

Ma nel nostro Paese c'è qualcosa di ancora più prezioso, che è quel perfetto equilibrio che nel tempo si

il disegno di legge sul consumo del suolo. Intanto ricordiamo che la legge sul sistema delle aree naturali protette del nostro Paese ha costituito un argine fondamentale al consumo del suolo e alla distruzione dei paesaggi più pregiati, custodendo un patrimonio di risorse ambientali insostituibile, ancora più prezioso nei tempi in cui viviamo, caratterizzati dai cambiamenti climatici

Questo sistema ha ottenuto successi indubbi, e non solo nella tutela degli *habitat* naturali e della biodiversità, che ho ricordato in precedenza, e nella conservazione della fauna e delle specie vegetali.

alla riscoperta e alla tutela della biodiversità agricola, allo sviluppo della agricoltura biologica. Il sistema delle aree protette, previsto nella citata legge, ha tolto dalla marginalità numerosi territori interni che, altrimenti, non avrebbero avuto alcuna alternativa all'abbandono. A fronte di questi contributi così importanti

essere superati i problemi che nel tempo si sono manifestati, possano essere implementate le risorse e il personale e si possa quindi mettere a disposizione, ancora di più,

sia assolutamente insufficiente nel merito e, per certi versi - e su questi punti mi soffermerò - anche controproducente. L'intervento del senatore D'Alì è stata - così l'ho definito - la voce dell'innocenza, se la vogliamo dire così, quella che svela anche alcuni scopi non proprio nobilissimi, almeno dal nostro punto di vista, che sono alla base del tentativo di rimettere mano alla legge quadro. Quando dico controproducenti individuo alcune aree critiche del testo che è arrivato in Assemblea. Innanzi tutto, mi riferisco alla *governance*, che è la questione più delicata e su cui si doveva intervenire per mettere in campo tutti gli strumenti per una *governance* di altissima qualità, in cui soprattutto gli interessi generali - sono quelli della gestione delle aree protette a scopi soprattutto di conservazione e di allargamento del sistema stesso

la giustissima dialettica - può produrre anche risultati importanti - tra la comunità del parco e gli enti gestori, per cui magari avremmo visto un sistema che rafforzava

avviene anche in assenza di una chiara definizione delle competenze specifiche che dovrebbero caratterizzare il profilo dei presidenti e dei membri del consiglio direttivo. In questo testo

è necessario - e abbiamo presentato alcuni emendamenti in merito - assicurare un equilibrio negli organi di governo tra i membri designati della comunità del parco e dei Comuni e la rappresentanza del mondo scientifico e associativo e, quindi, delineare con chiarezza le irrinunciabili competenze competenze in materia di conservazione della natura, di gestione delle aree protette, di tutela dei beni culturali e di economia dei beni ambientali sia del presidente che dei consiglieri.

in modo tale da eliminare qualsiasi possibilità di pressione sul parco che magari non ha altre risorse, quando devono essere rilasciate autorizzazioni di ogni genere.

strumenti molto più adeguati - a nostro avviso - per dotare il sistema dei parchi di una vera possibilità di finanziamento. L'altra questione da

perché ogni volta che la pronunciamo c'è sempre qualcosa di sbagliato che peggiora la situazione. Anche qui, con la riforma, dobbiamo mettere finalmente in grado i parchi di espandersi e di rilanciare il sistema. Bisogna mettere in campo personale adeguato, direzione e piante organiche.

il proprio direttore a prescindere dalle competenze, che saranno solo di natura amministrativa. Invece, occorrono competenze specifiche in un campo che non è come altri campi della pubblica amministrazione, perché riguarda la gestione delle aree protette. Arriviamo poi alla questione della gestione della fauna.

del silenzio-assenso in caso di mancanza di approvazione dei consigli regionali. Ci sono poi molte altre questioni, sulle quali noi abbiamo presentato anche emendamenti che potrebbero permetterci, alla fine, di sistemare

tutti gli strumenti per rilanciare il sistema, eliminando gli aspetti che ho indicato anche sommariamente e che rappresentano un elemento negativo e controproducente. Dobbiamo rilanciare i parchi e non affossarli, magari legandoli a logiche politicistiche e di interessi locali. La prima vocazione, la *mission* dei parchi è la conservazione e la tutela della biodiversità. Su questo si crea buona economia, su questo si crea occupazione. Ma oggi la

legge al nostro esame intende aggiornare la legge quadro sulle aree protette dopo venticinque anni dalla sua entrata in vigore e ci prospetta numerose modifiche. La brevità del tempo a disposizione mi consente di intervenire solo su qualche punto che ritengo importante per conferire al lavoro svolto in Commissione la necessaria completezza. Concordo pienamente con l'orientamento del disegno di legge di rafforzare l'azione di sviluppo dell'area naturale protetta. Concordo, cioè, con la necessità di garantire la tutela della biodiversità, del paesaggio, della flora e della fauna e, allo stesso tempo, lo sviluppo economico attraverso azioni di snellimento normativo nell'attività delle aree;

al mantenimento dell'attività umana nei territori di competenza, in generale periferici e interni. Proprio a questo proposito, in relazione all'esigenza di promozione economica e sociale, ritengo necessario che le nomine nel consiglio direttivo prevedano il coinvolgimento di esperti del settore turistico e del *marketing*, le cui competenze possono contribuire al rilancio dell'auspicabile sviluppo turistico ed economico dei territori interessati. Evidenzio che, se vi sarà la volontà in questa direzione, sarà possibile intervenire in sede di approvazione degli emendamenti. Un altro punto riguarda la nomina del presidente (articolo 4, comma 4). A mio avviso, nell'attuale formulazione permane una criticità che, peraltro, può essere anch'essa superata in sede di approvazione degli emendamenti. Mi riferisco alle forme di intesa tra Ministero e Regione. È preferibile fissare un termine entro il quale ottenere l'intesa, piuttosto che prospettare una modalità attraverso la quale, di fatto, escludere le Regioni non allineate Questa previsione rappresenta più un ostacolo che non una soluzione alla scelta condivisa del presidente dell'area protetta. A mio modo di vedere, ne va dell'autorevolezza del principale organo dell'ente. In merito, poi, all'articolo 5, permane una criticità laddove si riconosce alla federazione dei parchi la titolarità esclusiva della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti gestori. A nostro avviso, qualora si volesse procedere in tal senso, sarebbe necessario richiedere precisi requisiti utili ad assicurare principi di funzionamento dell'associazione ispirati a norme di trasparenza, universalità di accesso e garanzia di rappresentanza. Con modesto sforzo segnalo al relatore che, anche in questo caso, insieme al Governo potrà dare il via libera alle necessarie integrazioni, in particolare agli emendamenti che abbiamo proposto in merito.

Nel merito, va segnalato che la modalità dei pagamenti da parte di sistemi e impianti collocati entro il perimetro dei parchi assume al momento una quantificazione provvisoria. Auspico che tale provvisorietà possa a breve essere superata attraverso la necessaria interlocuzione tra Ministeri e portatori di interessi, tesa a definire l'effettiva sostenibilità dei pagamenti di cui si tratta. Segnalo al relatore la necessità di inserire anche il Ministero dello sviluppo economico nel novero dei Ministeri chiamati ad esprimersi, proprio per non far mancare all'approfondimento un apporto importante relativo ai settori della produzione e trasmissione di energia e alle attività economiche collocate all'interno del parco. Aggiungo, rimanendo in tema di PSEA, che non ho apprezzato il reinserimento all'ultimo momento dell'articolo 26, «Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici». La delega precedente è spirata senza aver fornito risultati apprezzabili; ma proprio questo è il sintomo di un'incertezza della materia, che andrebbe approfondita senza accelerazioni incomprensibili e con la necessaria dose di buon senso e aderenza alla realtà. Va ribadito qui quanto già espresso in sede di discussione sul collegato ambientale: la complessità della materia richiede un'analisi parlamentare specifica, al fine di fornire un quadro di riferimento esaustivo, completo di definizioni e di indicazioni operative scrupolose e dettagliate, con lo scopo di evitare l'insorgere di prevedibili contenziosi generati da indeterminatezza della previsione. A mio avviso, relatore e Governo meglio farebbero a riconsiderare l'articolo 26 e ad affrontare i contenuti degli PSEA in uno specifico Fra l'altro, non vorrei che l'esito finale della delega dell'articolo 26, vista la difficoltà ad operare adeguatamente, finisse con l'orientarsi sull'esistente (mi esprimo così), andando infine ad interessare canoni e sovracanoni idrici attualmente nella disponibilità di Regioni, Province e Comuni, compromettendo un sistema che funziona con efficacia sin dal testo unico delle acque del 1933 e che fornisce significative risorse ai territori ai territori interessati, senza bisogno di sovrastrutture centralistiche, costose e ovviamente contrarie alla sussidiarietà.

e dei criteri che le definiscono quali soggetti aventi carattere nazionale. La norma, così come impostata, sembra più escludere che facilitare la partecipazione, quando si prevede che le associazioni di protezione ambientale assumano carattere nazionale se presenti in almeno dieci Regioni: si pone un limite notevole, che non tiene conto delle singolarità e delle peculiarità che caratterizzano alcuni territori. A mio avviso, la soglia va ridotta proprio per permettere il riconoscimento della specificità dei territori, anche in relazione a particolari aspetti ambientali, paesaggistici e culturali tipici di aree di ridotta dimensione. Infine, in merito al tema delle aree contigue osservo che permane incertezza di trattazione. È necessario fare massima chiarezza di competenze e di intervento da parte dell'area protetta, in modo da evitare che esse vengano utilizzate come veri e propri strumenti impropri di espansione - lasciatemi dire così - non prevista e non programmata dell'area naturale,

ancora una volta quest'Assemblea è chiamata a discutere su un'importante legge, volta soprattutto a fornire alle aree protette nuovi strumenti per la tutela della biodiversità e la conservazione degli *habitat* naturali. È emblematico che il Senato della Repubblica si sia reso protagonista di un'importante stagione di riforme, soprattutto in campo ambientale. Basti pensare ai ventuno anni per l'approvazione della legge sugli ecoreati, otto anni per quella di riforma delle agenzie ambientali e ai sette anni per portare la discussione di questo provvedimento in questo consesso. Aggiornare la legge quadro delle aree protette, la n. 394 del 1991, rappresenta per noi la consapevolezza che i parchi italiani devono essere messi nella condizione di svolgere al meglio la loro funzione di conservazione del patrimonio naturale e della biodiversità, e la certezza che, in una concezione moderna della conservazione, nelle aree protette si possano creare nuove opportunità di sviluppo economico basato sulla identità e sulla qualità dei territori.

un traguardo notevole e non scontato, cui la politica deve restituire il giusto valore e la necessaria attenzione. La gravità dei danni causati dai cambiamenti climatici è sotto gli occhi di tutti nonché la perdita costante di biodiversità; la scorsa settimana abbiamo ratificato proprio in quest'Aula l'Accordo di Parigi per la riduzione dei gas climalteranti, assumendoci l'impegno di portare avanti azioni che ci permettano di centrare l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto della soglia dei due gradi. Uno dei modi per raggiungere questi importanti obiettivi è sicuramente la valorizzazione del ruolo delle aree protette, che oltre ad essere il mezzo principale per aumentare l'azione di conservazione e tutela dei nostri preziosissimi *habitat*, deve diventare per la coscienza collettiva lo strumento in grado di migliorare le nostre condizioni di vita, nonché un reale gesto di solidarietà generazionale. Non più la campana di vetro entro cui chiudere una porzione del nostro territorio, un qualcosa di inaccessibile: i parchi devono aprirsi alle comunità locali, devono coinvolgerle nella loro azione di conservazione e salvaguardia, con l'obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità anche alle aree limitrofe. Auspico che i parchi possano al più presto assumere il ruolo di soggetti istituzionali promotori di sviluppo locale e di volano per l'economia del territorio in cui ricadono. Sicuramente per adempiere al meglio a questi nuovi compiti, gli organi dell'Ente parco hanno bisogno di avere più potere e, insieme, di accedere a procedure decisionali più semplici e veloci. Tra gli aspetti più innovativi e significativi contenuti nel disegno di legge vorrei segnalare: il ricollegamento tra la Rete Natura 2000 e il sistema delle aree protette ai fini della conservazione della biodiversità (articolo 1); l'affidamento all'Ente parco della gestione delle aree della Rete Natura 2000 sia quando siano comprese nel territorio di parchi, riserve e aree marine protette sia, ove possibile, quando siano esterne a esso aver dato un ruolo determinante all'ISPRA come strumento tecnico scientifico per le aree protette (articolo 1); aver collegato le aree marine protette alle aree protette, con l'introduzione del parco nazionale con estensione a mare: l'estensione a mare ricomprende anche le aree marine protette contigue al parco terrestre, comprese le zone che non sono aree marine protette aver fissato le scadenze certe per la nomina del presidente dei parchi nazionali (articolo 4), per l'approvazione del piano del parco e del regolamento (articolo 5), per il rilascio di pareri, intese, pronunce; aver finalmente sancito l'incompatibilità del presidente con incarichi elettivi e con incarichi nella pubblica amministrazione aver abolito l'obsoleto albo dei direttori dei parchi, introdotto un concorso pubblico per la loro designazione, richiedendo più qualifiche e titoli l'attribuzione di maggiori poteri al presidente, che non solo coordina l'attività dell'ente ma esercita anche le funzioni di indirizzo e programmazione, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica del loro raggiungimento (articolo l'indicazione delle aree contigue nel piano del parco, d'intesa con le Regioni e non più su iniziativa di queste e una regolamentazione dell'attività venatoria in tali aree più chiara rispetto a quella vigente (articolo l'attribuzione agli Enti parco di competenze in materia di autorizzazione paesaggistica (articolo 22); il superamento del silenzio assenso nella concessione dei nulla osta (articolo l'unificazione dei piani (piano del parco e piano pluriennale economico e sociale) (articolo 5); la disciplina della gestione della fauna, che sviluppa e chiarisce principi presenti nella normativa vigente la concessione gratuita dei beni demaniali agli enti gestori delle aree protette, dai quali pertanto questi possono trarre anche risorse finanziarie, nonché di quelli sottratti alle mafie; sempre per il recupero di risorse l'aver introdotto il pagamento dei servizi ecosistemici; l'aumento, in generale del 100 per cento delle sanzioni pecuniarie e maggiore incisività della confisca dei beni (articolo 17); l'istituzione di nuovi parchi nazionali. Cambiare per migliorare era importante, ma non facile, perché, come ricordava il collega Caleo, bisognava in primo luogo affrontare gli scetticismi e con onestà intellettuale mettere in luce le parti della legge che non funzionavano. Ritengo che il lavoro condotto in questi mesi in Commissione sia un buon lavoro, che consentirà finalmente alle nostre aree protette di essere percepite come un'opportunità, come un fiore all'occhiello dalle comunità che le abitano. Un tema purtroppo ancora oggi non risolto è quello delle risorse. Senza il contributo dello Stato i parchi nazionali italiani difficilmente avranno la forza per impostare un percorso di rilancio di un modello di sviluppo locale che sia sostenibile e realmente competitivo. Il Parlamento sta facendo e farà la sua parte, ma ora il Governo può fare di più, anche a partire dalla prossima legge di stabilità, stanziando maggiori risorse per la salvaguardia del nostro inestimabile patrimonio di biodiversità.

Non furono proposte dal Governo, ma nacquero perché nel Paese si era sviluppata, negli anni precedenti, una discussione alla quale avevano apportato un contributo molto importante tante associazioni ambientaliste e tanti esponenti del mondo della ricerca e delle università, il mondo che faceva riferimento alla politica. Anche la politica e i partiti si interessarono in quegli anni all'ambiente e ai parchi; c'è stato proprio un cambio di passo, anche culturale. Nel 1991 il Parlamento percepì questa mutazione, anche grazie al contributo di intellettuali molto importanti che nel nostro Paese hanno fatto la storia

sei parchi regionali, sia costieri che dell'entroterra. Ho fatto questa premessa per dire che mettiamo mano

alcune correzioni che vanno a interagire con alcuni *vulnus* che si sono palesati in questi venticinque anni. Senza snaturare la struttura cercato d'introdurre elementi che potessero far ripartire con più forza, anche con entusiasmo, un sistema che si era un po' affaticato, con il rischio di afflosciarsi su se stesso. Era quindi un'operazione che andava compiuta con grande attenzione; credo inoltre che le leggi - me lo insegnate, colleghi - sono tutte migliorabili, però in quel momento noi avevamo di fronte un bivio che ci ha portato a fare delle scelte che sicuramente non stravolgono la struttura ma la rendono più forte, più trasparente, più efficace, dando un segnale di attenzione a un mondo che aveva determinate aspettative. Partendo da questi presupposti credo quindi che il lavoro

senza snaturare il significato del testo unico presentato, una valutazione positiva di alcuni emendamenti sicuramente (anche questa notte) cercherò di farla. In questo percorso c'è stata un'interlocuzione anche con il mondo ambientalista. Nella relazione introduttiva ho parlato di una interlocuzione, di un rapporto, di un dialogo con il mondo dei parchi,

quando si andava a parlare dei parchi si rischiava l'assedio: non eravamo accolti con le fanfare e con la musica sinfonica, bensì con grande scetticismo.

le associazioni di categoria agricole, gli operatori turistici e gli artigiani passare in questo ventennio da uno scetticismo e da un ostracismo molto importanti a una condivisione, ad un apprezzamento, al punto che adesso sono proprio i territori stessi e le comunità locali a chiedere di inserire pezzi di territorio all'interno dell'area protetta. protetta. È una soddisfazione personale, ma penso che sia soprattutto una maturazione dal punto di vista culturale e politico che bisogna cogliere come rappresentanti degli italiani nel Parlamento; abbiamo cercato di considerare questo aspetto ed abbiamo anche cercato di introdurre le correzioni che

delle lunghissime fasi in cui non c'è una direzione politica autorevole supportata da un'intesa tra Governo, Regioni e territorio. Abbiamo previsto tempi stretti, colleghi, perché pensavamo e pensiamo tuttora di dare la possibilità al Ministro di decidere, cercando l'intesa su una terna. Forse Forse non ci ricordiamo molto bene la legge n. 394 originaria, ma in tale proposta di modifica il profilo del presidente è molto definito definito e viene definito da particolari competenze che prima non aveva. Adesso invece individuiamo caratteristiche legate alla professionalità, alla competenza e alla gestione

mettere assieme e cercare di far dialogare una visione centralistica, ministeriale, con una visione locale: i parchi, se non riescono ad uscire dai propri confini, rischiano veramente di morire. Noi dobbiamo valorizzare molto di più e meglio non bisogna vedere il protagonismo delle comunità locali come un'invadenza, un'ingerenza rispetto a prerogative che deve avere lo Stato. Trovare il giusto equilibrio tra un'azione importante, un'impronta programmatica del Ministero e un sano protagonismo locale, credo non disturbi troppo la legge, a tal punto che

attraverso un albo che è fermo da trent'anni, dove c'è anche una presenza, una rappresentanza di ultracinquantenni. Credo sia importante dare un segnale anche ai giovani, in termini di selezione di capacità e di competenza che devono mettere a disposizione di questo Paese. Ho conosciuto in tanti anni giovanissimi preparati, laureati nelle più disparate discipline, non solo ricercatori laureati in scienze naturali.

come accaduto in questi anni, una sovrintendenza. Il direttore era vissuto come una sovrintendenza: il sovrintendente del Ministero presso le comunità locali. Abbiamo cercato di superare anche questo aspetto. Ho sentito parlare molto, anche in articoli sui giornali, del fatto che manca un orizzonte strategico alla nuova fase dei parchi e delle aree protette

stabilito per legge, di sostenere tutte quelle attività di ricerca, di monitoraggio, di programmazione e di pianificazione che i parchi vorranno mettere in campo.

importante verificare la fecondità dell'azione programmatoria di un parco, per fare in modo che esso non sia un elemento isolato.

parco potrà però produrre anche altri livelli di programmazione, che non sono solo legati all'attività venatoria, per quanto riguarda l'agricoltura, la caccia, la pesca, il turismo

di come il parco possa dare una mano, non solo per il rilancio del nostro entroterra, non solo per quanto riguarda il contrasto alla migrazione dei giovani, soprattutto dall'entroterra alla costa, per eliminare tutte le storture che portano ad un decadimento del territorio e alla difficoltà nel contenere il dissesto idrogeologico. c'è stata la volontà di far diventare il parco uno degli elementi centrali per il rilancio del territorio; a maggior ragione, Presidente, credo che ciò sia importante anche nella fase di ricostruzione. amministratori attenti, presidenti attenti, parlamentari attenti al territorio; si può prendere spunto da una storia triste del nostro Paese per dare l'immagine di un'Italia che vuole ripartire dalle sue bellezze più importanti, dalle sue emergenze storico-ambientali straordinarie. I parchi servono anche a questo.

Signora Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame rappresenta un importante strumento di valorizzazione del patrimonio ambientale e nella tutela delle risorse naturali del nostro Paese. Il Parlamento ha approvato, in questi due anni, un mosaico di riforme ambientali imprescindibili per un Paese come l'Italia, che guarda al futuro pensando all'economia verde come vero motore dello sviluppo. Il primo tassello - voglio ricordarlo - è stata la legge sugli ecoreati, con cui abbiamo introdotto certezze attese da anni su attività illegali come l'inquinamento e il disastro ambientale, il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività. A seguire, il collegato ambientale, una vera e propria

Tutte norme perfettamente coerenti con l'impegno preso alla COP21 di Parigi e con il modello di sviluppo dell'economia circolare proposto dall'Europa. Non voglio dimenticare la riforma delle agenzie ambientali, un altro tassello fondamentale che ci permette di costruire un sistema credibile e univoco in materia di controlli che dia certezze ai nostri figli, ma

Questa legge quadro - voglio ricordarlo - ha consentito l'affermazione di un sistema forte e coordinato per la tutela del patrimonio naturalistico e ambientale italiano. Come ha sottolineato la senatrice Puppato, si tratta di una legge straordinaria per l'epoca in cui è stata emanata. Oggi però si sente la necessità - come hanno detto molti onorevoli senatori - di rivederla, anche a fronte della mutata sensibilità

di una legge cornice che riscriva la *governance* in un'ottica attuale, che riveda le modalità procedurali, le finalità, le competenze funzionali, ma anche le regole per l'assetto del territorio. Oggi lo scenario politico, economico e sociale è fortemente trasformato e richiede un aggiornamento complessivo, che consenta alle aree protette, da una parte, di svolgere il ruolo che a loro naturalmente compete per la protezione dell'ambiente e della biodiversità, dall'altra, di rivederne quelle previsioni che hanno presentato aspetti di criticità nella loro applicazione. La *ratio* di questa legge non è di riaffermare il ruolo dei parchi italiani, che ormai è ampiamente riconosciuto, ma creare le condizioni affinché essi possano assolvere al meglio alle loro funzioni, che sono la tutela e l'accrescimento della biodiversità; l'educazione alla sostenibilità, la valorizzazione dei territori e delle economie locali, come ha sostenuto poc'anzi il senatore Caleo. Voglio sottolineare che il sistema delle aree protette tocca, con intensità differenti, oltre la metà dei Comuni italiani, costituendo un'importante risorsa verde anche per le città. Siamo passati, come hanno sottolineato tanti onorevoli senatori, dal 3 al 10 per cento di territorio nazionale tutelato. I parchi, in quest'ottica, devono essere considerati una risorsa finalizzata a migliorare la qualità della vita dei cittadini mediante azioni che promuovano e sviluppino l'economia verde.

di beneficiare di finanziamenti aggiuntivi rispetto alle risorse concesse annualmente dal Ministero dell'ambiente a valere sui fondi del proprio bilancio. Il disegno di legge individua criteri sulla nomina e sullo *status* dei membri degli organi dell'ente in modo più coerente con le necessità di garantire l'integrazione tra le diverse competenze. Infatti viene assicurato che il 50 per cento dei membri del consiglio direttivo sia designato dalla comunità del parco, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa comunità del parco, mentre il restante 50 per cento viene scelto tra esperti in materia naturalistica e ambientale su designazione dei soggetti istituzionali indicati nella norma. Riprendo quanto detto dal senatore D'Alì: vi è un maggiore coinvolgimento degli enti locali. Viene inoltre istituito un comitato nazionale per le aree protette con funzioni consultive, che predispone, in particolare, l'elenco ufficiale delle aree naturali protette sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente e una relazione annuale sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti. Si riprendono una serie di semplificazioni procedimentali. In primo luogo, il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco, che assolve anche alla funzione di nulla osta paesaggistico. In secondo luogo, viene introdotta una procedimentalizzazione della formazione del piano del parco e del regolamento. il regolamento del parco sarà anche lo strumento di pianificazione nel quale dovranno essere definiti gli interventi di controllo della fauna selvatica ai fini di tutela della biodiversità, pur mantenendo comunque il divieto di attività venatoria all'interno del parco. Si procedimentalizza, inoltre, la fase di acquisizione dell'intesa ai fini della nomina del presidente. Si disciplina con una modalità diversa, che comunque garantisce l'espletamento di una procedura selettiva, la nomina del direttore del parco, eliminando l'albo dei direttori ma assicurando una coerente disciplina che, senza penalizzare le professionalità necessarie, apre ad un confronto competitivo senza possibilità di meccanismi di chiamata diretta e conformemente alle disposizioni sulla dirigenza pubblica e sull'anticorruzione. inoltre previste nuove norme in materia di riserve marine semplificando la precedente disciplina. Un'ulteriore novità è l'autofinanziamento. Nell'ottica di valorizzare una gestione degli Enti parco improntata ad un maggiore ricorso ai proventi a loro favore, in aggiunta ai finanziamenti che il Ministero dell'ambiente provvede annualmente a destinare agli Enti parco a valere dalle risorse del proprio bilancio, si prevede un contributo a carico di soggetti che pongono in essere nel territorio del parco e delle aree anche contigue attività potenzialmente o effettivamente impattanti per l'ambiente, da destinare al risanamento ambientale e alla conservazione del patrimonio del parco. Sono certa che il Ministero dell'ambiente, anche con il supporto di questa Assemblea, cercherà sempre di dare risposte concrete a tutti quei territori che chiederanno di essere affiancati nella tutela e valorizzazione delle risorse naturali che devono essere custodite. Nel provvedimento viene inoltre previsto il conferimento di alcune deleghe al Governo. In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che riforma l'assetto ordinamentale e organizzativo delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, istituendo il Parco del Delta del Po sulla base di una legge speciale che sarà adottata in coerenza ai criteri di delega. Questo, come hanno detto nel corso del loro intervento sia il senatore Dalla Zuanna che la senatrice Puppato, riveste un carattere di grande importanza perché incide su un bacino di popolazione rilevante con un patrimonio naturalistico di primissimo livello, che nel 2015 è stato inserito nel programma MAB UNESCO. Inoltre, ulteriore delega viene prevista per l'introduzione di un sistema di volontariato di volontariato di remunerazione dei servizi ecosistemici (PES), e questo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Mi auguro che il provvedimento in esame, come hanno auspicato il senatore Caleo e il senatore D'Alì, possa essere approvato in tempi brevi, per dare quelle risposte che il mondo dei parchi ci sta chiedendo da tempo. Vorrei in ultimo ringraziare la Commissione per l'egregio e proficuo lavoro svolto, in particolare il presidente Marinello, il consigliere De Salvo,

Una relazione così corposa ha evidentemente una ragione d'essere, che adesso cercherò di spiegare, allungandomi un po' per quanto riguarda gli aspetti rilevati nel corso di un paio di anni di lavoro e che hanno riguardato l'ascolto, lo studio e l'analisi di diversi attori tecnici, politici, magistratura, procure, associazioni e anche lavoratori. hanno reso evidente un quadro decisamente multiforme per questa Regione italiana, talvolta di rilievo assolutamente positivo, ma spesso evidenziando lacune, che abbiamo ritenuto doveroso esporre doviziosamente in questo ampio *excursus* contenuto nella corposa relazione, Va detto subito che leggendo le prime sette pagine si respira aria buona, per così dire. Siamo la prima Regione d'Italia per quanto attiene la raccolta differenziata, con il 64,6

una quantità di rifiuto ad abitante tra le più basse dell'intero panorama nazionale e valori *pro capite* quasi doppi rispetto alla media nazionale, relativamente alla raccolta organica.

particolarmente evoluti e responsabili, abbiano prodotto un sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti che è diventato riferimento europeo, una *best practice* europea. però non ha nulla a che vedere, come vedremo in corso di trattazione, con il modo in cui è stato gestito normalmente il rifiuto, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti speciali e industriali e i fanghi di depurazione nell'ambito della stessa medesima Regione del Veneto. Altri valori interessanti e positivi sono gli impianti. In Regione Veneto si può sicuramente parlare di sistema impiantistico dedicato alla valorizzazione e al recupero delle frazioni secche riciclabili, con oltre 1.100 impianti di selezione e recupero per 11 milioni di tonnellate di rifiuti trattati. Si tratta, quindi, di piattaforme in cui vengono trattati sia rifiuti raccolti in Veneto, sia rifiuti *extra* Veneto, soprattutto per la parte speciale, ma anche per la parte urbana. In particolare, vanno rilevate le situazioni relative

ora al tema del *business* dei rifiuti. Evidentemente, un'impiantistica di queste dimensioni può far parlare di una gestione relativa alla materia prima e seconda di un alto livello

possiamo leggere un inciso significativo: «il reato di cui all'articolo 260, nella realtà veneta, si è posto subito in modo particolare la maggior parte dei casi riguarda aziende di medie dimensioni, che lavorano e trattano regolarmente rifiuti. Nella prassi, spesso si verifica che le indagini sulle contravvenzioni pongono in evidenza che il fenomeno non è episodico, in quanto si è in presenza di situazioni reiterate, sistematiche, tanto che alla fine si può configurare l'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, quindi di attività organizzate continuative connotate da finalità di profitto.

una serie di comportamenti deviati rispetto alla struttura normativa e alle prescrizioni fissate in sede amministrativa. Accade, cioè, che l'impresa riceva rifiuti anche pericolosi, comunque non compresi nel codice CER per cui è autorizzata e provveda alla loro successiva miscelazione con i rifiuti per cui è autorizzata». grazie a pieghe dei controlli non particolarmente efficaci, si opera in maniera difforme da quella prevista, con distorsioni delle regole di mercato. Le pratiche più in uso che producono lo smaltimento illegale di consistenti quantitativi di rifiuti sono quelle del cosiddetto giro bolla, cioè dell'operazione, da effettuarsi evidentemente presso un impianto di stoccaggio, di sostituzione del documento di accompagnamento originario del rifiuto, riportando indicazioni false o di comodo, quindi con un codice CER immutato, al fine di poterne accelerare il recupero o lo smaltimento. Il miscuglio di rifiuti è dunque difficile da contestare e anche da controllare, atteso che le sue caratteristiche sono piuttosto indeterminate si diceva, difficili anche da caratterizzare mediante un'analisi rispetto al singolo rifiuto determinato da un processo produttivo ben preciso. Quindi, il trasporto di miscele di rifiuto,

per quanto riguarda una figura apicale, l'ingegnere Fabio Fior. Ci si stupirà, quando parliamo di un argomento di tanta rilevanza, che ci si appigli ad una singola identità. Ebbene, questa storia ha davvero dell'incredibile, perché la quantità di incarichi apicali che questo ingegner Fior ha avuto a partire dall'anno 2000 cessando solo nel 2014 è davvero incredibile. Nella lunga carriera ai vertici dell'amministrazione regionale 2014: dirigente apicale della direzione tutela ambiente, contestualmente vice presidente della commissione tecnica regionale per l'ambiente (CTRA), a partire dal 5 luglio 2002 e fino al 23 agosto 2010, vice presidente della commissione di valutazione di impatto ambientale, poi dirigente del settore energia, quindi, dal 1° aprile 2014, dirigente del settore del progetto integrato Fusina per la sezione Venezia,

quindi tutte le aziende che intendevano presentare richieste di autorizzazione dovevano transitare attraverso il suo ruolo dirigenziale. Ma a lui competevano anche le autorizzazioni integrate ambientali e infine e infine poteva eseguire anche l'attività di collaudo dei relativi impianti, visto che sostanzialmente qualche centinaio di autorizzazioni in tal senso gli sono state concesse nel corso di quindici anni da parte della Giunta regionale del Veneto. Ma non contento, grazie ad una legge unica in Italia, la legge n. 3 del 2000, che aveva istituito solo in Veneto la figura del terzo controllore per un piano di controllo...

Dicevo che ha costituito all'uopo una sfilza enorme di società prestanomi, che non sto qui ad elencare, e ha avuto una quantità impressionante di appoggi politici e tecnici. La sua figura ha intersecato il MOSE e il Consorzio Venezia; questa figura, insieme o forse connivente con le aziende che inizialmente hanno gestito la questione relativa alla gestione dei rifiuti nel Veneto, ha certamente portato ad una sorta di sorta di palude nell'ambito della gestione dei rifiuti, che ha evidenziato nel corso di questi anni molte lacune.

all'attenzione nazionale per una nube tossica che si è scatenata ed ha provocato la morte di quattro operai. Infatti questa azienda che era per l'appunto affiliata a questo sistema di opacità

posteriormente) che questo materiale in uscita era solo un quinto di quello in entrata.

dalla relazione sul SIN di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, approvata all'unanimità dalla Commissione di inchiesta sulle ecomafie lo scorso 14 luglio 2016, emerge chiaramente - come peraltro accaduto per la relazione sui poli chimici che la messa in sicurezza e la bonifica dei siti industriali contaminati comporta un'impellente necessità di intervento, sia per l'esigenza di eliminare le fonti di inquinamento al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, sia per permettere la reindustrializzazione di aree, così da assicurare lo sviluppo industriale del Paese, difendendo contemporaneamente l'esigenza di evitare l'ulteriore consumo di suolo agricolo. Il SIN di Bussi sul Tirino, istituito nel 2008, comprende i territori di 11 Comuni e si estende dal polo chimico ad aree limitrofe, passando attraverso le Gole di Popoli, lungo la Valle del Pescara, fino alla confluenza del fiume Orte, dove sono presenti impianti industriali dismessi. Si trova in una posizione estremamente critica, dove si concentra circa un terzo di tutte le acque dell'Abruzzo, con scorrimento sia superficiale (fiume Pescara e fiume Tirino, suo affluente) che sotterraneo e al confine (a proposito di parchi) tra il Parco nazionale Gran Sasso e il Parco nazionale Maiella Morrone. La contaminazione delle matrici ambientali deriva dalle attività industriali esercitate per oltre un secolo nel polo chimico,

che potrebbe auspicabilmente preludere al progressivo reinsediamento di nuove attività, ovviamente con produzioni a minore impatto ambientale nella medesima area, caratterizzata da posizionamento strategico ed esistenza di adeguate infrastrutture. La Commissione, in occasione degli approfondimenti, ha tuttavia rilevato molte criticità e ritardi nella gestione commissariale, peraltro cessata nello scorso mese di giugno. È da sottolineare come, nonostante il sito e la sua gestione commissariale, iniziata nel 2007, abbiano fruito, nel corso del tempo, di norme speciali, anche primarie, introdotte al fine di garantire al commissario risorse economiche e la prosecuzione del suo mandato, nonché di norme secondarie e provvedimenti amministrativi aventi la medesima finalità, l'efficacia del modello di gestione commissariale si è rivelata decisamente insufficiente, anzi, oserei dire fallimentare. Diversi i fattori critici emersi: la la molteplicità dei livelli istituzionali coinvolti; l'interesse non adeguatamente canalizzato degli enti locali; il ruolo della Regione Abruzzo come soggetto esponenzialmente presente e rappresentativo, ma senza competenza tipizzata; il rapporto di scarsa collaborazione tra commissario e altri soggetti, tra cui il Ministero; la sovrapposizione di competenze e la presenza pubblica in una logica più di metodo procedurale che di risultato. Criticità che hanno prodotto atteggiamenti talora attendisti delle aziende insediate nel sito, nonché l'arenarsi di provvedimenti amministrativi nel contenzioso giudiziario. La situazione si è poi evoluta in occasione dell'approvazione dell'ultima legge di stabilità, che ha previsto la chiusura della decennale gestione commissariale al 30 giugno del corrente anno, anche se la fase post-commissariale ancora ad oggi ha sortito effetti visibili. In concreto la situazione della contaminazione del sito risulta irrisolta e, anzi, si sovrappongono in maniera singolare attività di messa in sicurezza, di bonifica e anche di caratterizzazione relative a più aree del SIN, denunciando - e ahimè confermando - una storica disorganicità di intervento complessivo, con un variegato e lento procedere e una scarsità di risultati effettivi. Continua a preoccupare il potenziale impatto della contaminazione sulle popolazioni, ad oggi non efficacemente esplorato con indagini epidemiologiche la cui attuazione rimane assolutamente necessaria. Anche le attese delle comunità locali relative alle vicende giudiziarie in ordine all'individuazione di responsabilità che provocassero riflessi sulla gestione del sito sono andate purtroppo deluse. I processi per i delitti di avvelenamento di acque e di disastro innominato, infatti, dopo i proscioglimenti in primo grado e una pronuncia della Corte di cassazione è tornato in corte di assise di appello. La vicenda del SIN di Bussi sul Tirino è un'ulteriore conferma dei limiti delle gestioni straordinarie e dell'utilità della riconduzione delle attività di bonifica alle procedure e alle competenze ordinarie, purché esercitate attivamente e positivamente. In questo ambito è fondamentale che le conferenze dei servizi non devono essere intese come luogo paludoso di sedimentazione dei processi, bensì come modulo risolutivo per il sollecito e fattivo esame congiunto degli interessi coinvolti, tale da produrre un'accelerazione dei tempi del procedimento. Nonostante i diversi anni, risulta ancora necessario - ahimè e questo è grave denunciarlo - valutare correttamente quante risorse pubbliche si rendono ancora necessarie per completare le attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza e bonifica del SIN, valutazione resa problematica dalla pregressa disorganicità dell'intervento. Superata la gestione commissariale, la presenza del Ministero dell'ambiente ovviamente non potrà prescindere dall'impiego di queste risorse economiche per la bonifica dei siti inquinati. È chiaro che anche l'esclusione dei saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle risorse destinate agli enti locali per le bonifiche potrà costituire un sostegno concreto. Grazie. è oggetto di modifiche, osservazioni e interlocuzioni estenuanti da parte dei soggetti istituzionalmente coinvolti: sto parlando del Ministero dell'ambiente, della Regione Abruzzo e dei Comuni coinvolti. coinvolti. Queste incertezze allontanano la messa in sicurezza e la bonifica di questi siti di interesse nazionale. Mi avvio alle conclusioni, chiedendo ai colleghi dell'Assemblea di fare propria la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta e impegnare il Governo, per quanto di competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione, in raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, le Regioni e gli enti territoriali interessati.

In una prima parte della relazione si è trattato il tema in forma generale, poiché il modello di gestione siciliana è riproposto, con caratteristiche alquanto simili, in tutto il territorio: un sistema patologico, basato su una diffusa illegalità, che trae agio che trae agio dall'inefficienza sistemica dell'amministrazione pubblica, facilitata da una gestione emergenziale continua che è durata più di quindici anni. La prima dichiarazione di emergenza risale al 1999, quando si pensò di porre fine al modello di smaltimento basato sulle discariche (una per Comune). Eppure, ancora oggi, si smaltisce in discarica il 90 per cento dei rifiuti, non ovunque e non sempre trattati in modo conforme, con un 10 per cento di raccolta differenziata:

gestiti dalla ditta Tirreno Ambiente SpA, e nella discarica Catania, gestita dalla ditta sicula Trasporti Srl. I risultati dell'inchiesta ispettiva sono stati utilizzati dagli uffici della procura e hanno portato all'emanazione di provvedimenti cautelari personali e reali. È chiaro che il sistema discariche, con le continue emergenze, abbia favorito economicamente i gestori privati, anche a causa di una gestione pubblica quasi inesistente, tranne per quanto riguarda la discarica di Bellolampo a Palermo, che non rappresenta comunque un esempio positivo di gestione. Nel 2002 si decise di costruire quattro inceneritori e questa decisione compromise senz'altro lo sviluppo della raccolta differenziata. Nel contempo si decise la costituzione di ben 27 ATO, che hanno causato causato grandissime disfunzioni ed esautorato i Comuni delle proprie competenze, causando anche una notevole crisi finanziaria che si protrae fino ad oggi. La gestione è stata deficitaria e non trasparente, ma perlopiù perlopiù appare chiaro che si è trattato di uno strumento in mano alla politica locale per il controllo del consenso. Ad oggi sembra (ma non è certo saperlo) che il debito di questi enti sfiori i 2 miliardi di euro. Dopo quindici anni di commissariamento non si sono fatti passi in avanti; molti territori sono invasi dai rifiuti e si profila la soluzione non soluzione di portarli fuori Regione. Un risultato i provvedimenti emergenziali e derogatori lo hanno avuto: è stata la procedura d'infrazione europea per violazione di molti articoli della direttiva n. 98 del 2008 sui rifiuti. Ne è emersa una mancanza di volontà politica, un'incapacità gestionale e sicuramente la concussione. Non è stato portato avanti nessun processo pianificatorio, procedendo sempre per misure straordinarie senza nessuna prospettiva di sblocco all'orizzonte, neanche ad oggi, direi neanche con la nuova ordinanza regionale contingente ed urgente n. 5 del 7 giugno, che sostituisce gli ATO e le società di che impone ai Comuni l'utilizzo di discariche a centinaia di chilometri di distanza, con un gravissimo aggravio dei costi. Si tratta, dunque, di un ennesimo provvedimento in deroga alle direttive comunitarie in materia. Quindi, se è vero che il Ministero non ha concesso un nuovo commissariamento, di fatto ha concesso la possibilità di varare una nuova ordinanza contenente prescrizioni stringenti dettate dal Ministero, quindi cambia Si continua a trattare la raccolta, il trattamento, l'abbancamento, l'adeguamento dei piani regionali e l'impiantistica con provvedimenti derogatori che escludono e deresponsabilizzano gli enti locali.

che è stata allo studio della Commissione, dal bando per i quattro inceneritori, che è uno dei più recenti, e dalla verifica delle autorizzazioni per le discariche emergono una mancanza sistemica di controlli e una corruzione altamente ramificata in tutti i settori della politica, dell'amministrazione e delle professioni che generano introiti illegittimi illegali e quindi criminali. Il sistema delle maxidiscariche ha causato un elevato inquinamento delle aree limitrofe, che ha sollevato giustificati dubbi di illiceità sulle modalità con cui sono state rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali, ne è emersa la patologia di un'impropria commistione tra funzionari pubblici e imprese private: la stratificazione normativa e la macchinosa burocrazia facilitano il gioco di funzionari corrotti. È da segnalare come nelle inchieste sia risultato che medesime società operanti nel settore dei rifiuti, presenti in diverse inchieste giudiziarie, continuino ad operare nel settore in più parti d'Italia. L'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso, che controlla molto bene il territorio, ha reso possibile anche la realizzazione di una maglia fittissima di discariche abusive. Ma ciò non sarebbe mai stato possibile senza la mancanza assoluta di controllo da parte degli organi preposti. Questi ingenti quantitativi di rifiuti che girano in tutta la Sicilia fino ad arrivare ai siti non autorizzati non sono stati visti da nessuno. La magistratura in tutto questo fa attività di supplenza rispetto alla quasi totale insufficienza della pubblica amministrazione, e recentemente fa così anche l'ANAC; ma certo questa non può essere una soluzione. Chiediamo al Governo di fare propria questa relazione e di intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta e quindi di emettere provvedimenti atti a superare questi problemi. Avverto che le eventuali proposte di risoluzione ai documenti in esame potranno essere presentate entro la conclusione della discussione congiunta, che si svolgerà nella seduta di domani mattina.

Grazie.